la prima votazione, come consuetudine, attendo, perché ci sono senatori che stanno ritirando la tessera.

appoggiata)*. Colleghi, per cortesia, vi invito a prendere posto, onde evitare risse da stadio. Invito

di articolare diversamente il nostro calendario dei lavori, di concentrarci sui temi su cui è possibile trovare delle intese, per dare ai mercati il segnale che l'Italia, le sue istituzioni

almeno nel metodo, era stata raggiunta. Ma possibile che non si possa essere all'altezza della sfida che il nostro Paese sta affrontando? L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Il tema è molto interessante e di grande attualità, perché il mondo giuridico si interroga da diverso tempo sull'argomento. È giusto o no che per i delitti più gravi ed efferati, per i quali viene prevista quale pena massima comminabile quella dell'ergastolo cioè «fine pena mai», com'è scritto nei documenti carcerari - sia stabilito un automatismo che, per la sola scelta del rito, porterà il beneficio di una riduzione di pena dall'ergastolo a 30 anni?

Con una decisione improvvisa, quanto inopportuna, la Commissione giustizia ha deciso di sopprimere gli articoli più significativi del disegno

pena, dedicandosi ad inserire una questione tutta diversa e completamente eccentrica rispetto al tema, cioè l'ampiezza del diritto alla prova. decisione estemporanea ed inopportuna, perché qui si sta parlando di altro: si sta discutendo della compatibilità di un rito abbreviato, introdotto con finalità deflattive, con delitti gravi che la pubblica opinione vorrebbe puniti senza troppo sconti. Invece, accanto a questo tema, si viene ad introdurre una questione che nulla c'entra, perché riguarda essenzialmente il dibattimento, cioè un'altra fase del procedimento penale. Viene infatti modificato l'articolo 190 del codice di procedura penale sul diritto alla prova; verrebbero sostituiti due commi, che praticamente ampliano i diritti dell'imputato, testualmente - «di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni mezzo di prova a suo favore». Ciò avviene senza alcun filtro, senza alcuna possibilità di selezione da parte del giudice. Mi spiego meglio. Se un difensore ha un interesse processuale ad allungare i tempi, magari per favorire la prescrizione del processo, e deposita una lunga lista testimoniale, che di fatto paralizza l'attività dibattimentale, può farlo. Per questo i *media* hanno parlato di «processo lungo». È vero, un problema esiste sul tema del diritto alla prova, e bisognerà trovare un meccanismo che tolga i difensori dalla preoccupazione di una decisione magari

celebrazione in tempi ragionevoli di molti processi, che invece potrebbero essere definiti molto più celermente, garantendo ugualmente la parte e quindi la difesa. È evidente che ci troviamo di fronte, di nuovo, ad una norma *ad personam*. Sul problema del giudizio abbreviato per i delitti più gravi anche il Partito Democratico ha presentato in Parlamento alcuni disegni di legge, nei quali viene stabilito che ai reati che prevedono la pena dell'ergastolo non si possa applicare la riduzione di pena prevista dalla scelta del giudizio abbreviato: quello del collega senatore Maritati è stato firmato anche da molti altri componenti della Commissione giustizia del Senato, ma ricordo anche il disegno di legge a firma D'Ambrosio. In questi anni, abbiamo visto che spesso, quando viene commesso un omicidio, al processo viene comminata una pena che dall'opinione pubblica viene ritenuta non adeguata alla gravità del fatto. Spesso, come battuta, si sente dire che in galera non ci va più nessuno, neanche per l'omicidio. La riduzione della pena, dall'ergastolo a trent'anni di reclusione, per la sola scelta del rito, comporta che il riconoscimento di eventuali attenuanti generiche o specifiche ad un'azione delittuosa porti poi la pena sotto i vent'anni di reclusione, o ancora meno se vengono riconosciute altre circostanze. Poi, con la liberazione anticipata o altri benefici, che legittimamente con il buon comportamento detentivo il condannato può ottenere, dopo otto, dieci o dodici anni può lasciare il carcere per essere avviato ad una nuova fase di graduale reinserimento sociale. Ecco, questa avrebbe dovuto essere l'occasione per il legislatore di intervenire senza alcun costo, quindi senza necessità di copertura di bilancio, su un argomento delicato e importante, sul quale eravamo disposti a discutere in maniera costruttiva, ma senza inserire in questo disegno di legge norme che hanno tutt'altro fine e che per la loro consistenza allungherebbero significativamente la durata dei processi. Un'ultima considerazione politica: avevamo pensato che dopo le elezioni amministrative, dopo il *referendum*, dopo i sondaggi negativi e durante una crisi che sembra non trovi uno spiraglio di soluzione, dopo tutti i segnali che il Paese reale sta mandando alla politica, la maggioranza avesse abbandonato la via delle leggi *ad personam* e di una giustizia a misura dei problemi legali del *Premier*. A nulla è servito l'immane sforzo dell'opposizione

un contenuto non condiviso, al solo scopo di evitare che i mercati europei e italiani fossero sottoposti ad un nuovo assalto. Con questa nuova forzatura e con l'approvazione di questo disegno di legge dimostrate al Paese che non è cambiato nulla che la vostra prima preoccupazione era ed è ancora andare avanti a colpi di maggioranza con l'approvazione di leggi che non migliorano la qualità della vita degli italiani, non aiutano il sistema giudiziario né sostengono il lavoro, le imprese e neppure l'economia. Sono le solite leggi *ad personam*, e null'altro. Eppure, anche solo da un punto di vista tattico o politico, a mio modesto parere avete perso un'occasione politica per risintonizzarvi con il Paese: e di questo l'opposizione dovrebbe ringraziare, se non ci fosse la preoccupazione per l'interesse generale del Paese, che fuori da quest'Aula continua a chiedere alle istituzioni e al Governo le riforme necessarie.

*(PD)*. Signora Presidente, c'è da chiedersi veramente che Paese sia il nostro.

per quanto riguarda i reati di competenza della corte d'assise spetta alla competenza della corte d'assise. In verità non si riesce a capire se ci sia un qualche legame tra il Governo che è il Governo che è presente alla Camera e il Governo che prepara questo disegno di legge al Ministero della giustizia e poi lo presenta al Senato.

nel codice del 1988, entrato in vigore nel 1989, si prevedeva che il giudizio abbreviato si applicasse anche ai reati puniti con l'ergastolo. Dopodiché, nel 1991, intervenne una sentenza della Corte costituzionale perché giustamente lasciava perplessi che ciò fosse possibile, e

Devo dire che a questo punto l'iniziativa della Lega alla Camera dei deputati trovava una spiegazione molto precisa nel fatto che, per delitti gravissimi,

sui riti alternativi si è sempre discusso, ma lo si è fatto soprattutto in relazione all'incidenza sui tempi di definizione dei processi. Quando entrò in vigore il nuovo codice di procedura penale, si capì immediatamente che si trattava di un processo difficile da far funzionare, che avrebbe richiesto tempi davvero quanto la prova veniva raccolta in dibattimento. Allora si pensò di fare ricorso ai riti alternativi per evitare

Poiché non funzionavano questi riti alternativi, si è intervenuti nel 1999 con la legge Carotti modificando l'abbreviato, facendolo diventare un diritto dell'imputato ad avere una riduzione di pena chiedendo il rito abbreviato e introducendo quindi una forma di nuovo giudizio

Anche questo esperimento è fallito completamente, perché, stando alle statistiche, i riti abbreviati non sono aumentati. Allo stesso modo si è agito con

Il senatore Mugnai faceva riferimento all'obbligo di raccogliere in sede penale anche le prove inerenti al al risarcimento dei danni. Ma vi rendete conto di quel che succede invece in concreto? Mai che venga stabilito in sede penale il risarcimento dei danni! Ma attenzione, quando Ma attenzione, quando noi ricorriamo all'applicazione della pena su richiesta delle parti, quella sentenza viene equiparata alla sentenza di condanna, ma non fa stato nel processo civile. Voi dite che i processi civili ed

era previsto un sistema nel codice, perché quel che si dimentica è che se è vero che era contemplata l'ammissione delle prove, tuttavia le relative ordinanze potevano essere sempre modificate. Non solo, noi abbiamo anche l'appello, in cui si possono ammettere nuove prove

ben descritto da tutti i colleghi che mi hanno preceduto, per allungare ancor di più i tempi di questo processo? E allo stesso tempo, in Commissione c'è un disegno di legge che prevede, per gli incensurati,

riduciamo i tempi di prescrizione, il che vuol dire che in questo modo non renderemo giustizia alla gente e non avremo mai investimenti di imprese straniere in Italia. Signora Presidente, rilevo preliminarmente che quando discutiamo di problemi attinenti alla giustizia, soprattutto in questa legislatura, l'Aula del Senato si svuota, soprattutto nei banchi della maggioranza. Credo che molti colleghi della maggioranza preferiscano rifugiarsi nella *buvette*, perché hanno vergogna. Io questo lo percepisco, lo sento. Il concetto che sto esprimendo adesso non vuole essere provocatorio, perché coloro i quali si vergognano, e lo dicono in discorsi a quattr'occhi, perlomeno fanno salva la dignità, si sottraggono dal mettere la testa sotto la sabbia per non guardare quel che stiamo facendo. Io penso si debba ragionare con serenità,

ha tentato, ed in parte ci è riuscito, di ridare un certo senso di dignità a tutti i colleghi di Gruppo, che poi gli hanno battuto le mani, dicendo cose peraltro abbastanza inesatte (lo vedremo tra poco). Ma l'enfasi di Mugnai è proprio legata a questo stato di prostrazione in cui voi ragionevolmente state cadendo, per questo tipo di norme che voi irresponsabilmente state varando a danno del Paese. È stato introdotto nella Costituzione il principio del giusto processo. Certo, noi la leggiamo la Costituzione, la conosciamo, e nel principio del giusto processo non c'è soltanto la facoltà per l'imputato di interrogare o far interrogare: c'è innanzitutto

sono molto impegnati e tengono molto ad affermare determinati principi: con il senatore Mazzatorta ho parlato di questo disegno di legge lui, inizialmente diffidente, si è poi reso conto che quello a mia firma era identico nella sostanza, e che potevamo marciare insieme. Allora, io chiedo ai colleghi della Lega: che cosa è accaduto per cui questo disegno di legge è stato stravolto, e sotto i vostri occhi, o con il vostro consenso - spero proprio di no è stato introdotto qualcosa che va in una direzione diametralmente opposta a quella del principio costituzionale del giusto e ragionevole processo? Non c'è soltanto il diritto alla difesa, sacrosanto diritto alla difesa, nella nostra Costituzione: ci sono interessi e valori parimenti da tutelare, quali quello della difesa sociale il diritto a conoscere la verità dei fatti. In questi giorni abbiamo affrontato temi delicati che riguardavano uno di noi, e voi da quei banchi avete gridato. Ricordo qualcuno di voi che gridava e leggeva le intercettazioni telefoniche. Siamo nella fase preliminare: quando sapremo la verità su quei fatti? Quando sapremo la verità su altri fatti di cui oggi parlano i giornali, e parleranno, di questi scandali? Continueremo a parlare solo della fase dell'indagine preliminare? catture, di queste catture che vengono emesse in maniera facile e superficiale da pubblici ministeri che sono giudicati oggi pazzi, domani, o nello stesso tempo,

a quelli relativi ai tempi biblici dei processi, che non vengono a conclusione, per cui noi discutiamo, ci confrontiamo, ci dividiamo ma non sapremo mai la verità sui fatti su cui ci siamo scontrando. sono passati tre anni e vi abbiamo proposto riforme sagge, riforme che non prendono le mosse da un punto di vista di sinistra o politicamente classificabile, ma che necessarie al buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Avete sistematicamente chiuso gli occhi, vi siete messi a pensare ad altro e avete imposto con la sola forza dei numeri, senza mai ragionare, una serie di norme, alcune delle quali neutralizzate dalla Corte costituzionale: norme utili solo a salvare o a strappare dal giudizio dei tribunali di questa Repubblica il Capo del vostro Governo, il vostro capo di partito. Questo non rende onore alla storia vostra, alla storia dell'Italia, e ha determinato un blocco e una regressione costante del nostro Paese sul piano della giustizia e dei valori costituzionali, sul piano dell'uguaglianza e del rispetto della persona. persona. E questa legge che vi accingete a votare, la gran parte di voi non l'ha letta, non vuole comprendere di che cosa stiamo trattando e preferisce star fuori dall'Aula. Chi invece si rende conto di tutto questo non dice nulla: ha parlato solo Mugnai, e tra poco dirò che cosa ha detto di inesatto. Viene introdotto - a fianco del rito abbreviato, che ritengo sia giusto non debba essere concesso a chi si rende responsabile di gravissimi delitti - un sistema di assunzione delle prove che sconvolge il nostro sistema.

Qual è l'esigenza concreta da cui siete partiti? Quali sono i fatti, i processi all'interno dei quali è stata avvertita l'esigenza di avere un numero illimitato di testimoni, mentre ci sarebbe stato un intervento irrazionale di esclusione da parte dei magistrati? Non abbiamo notizia di tutto questo. Improvvisamente si prende questa previsione costituzionale, la si estrapola, la si inserisce in un contesto che non conosce l'istituto dell'interrogatorio diretto e crea e creerà - se non sarà accompagnato da una riforma complessiva e organica, sulla quale siamo pronti ad intervenire - danni enormi. Il mafioso, lo stupratore, il rapinatore, l'estorsore, il criminale - comunque pericoloso - interrogherà, guardandola negli occhi, la sua vittima, interrogherà i testimoni (quando ci sono, e naturalmente ve ne saranno sempre di meno) che lo hanno accusato o che riferiscono di circostanze e condizioni a suo carico. lo recita la Costituzione: certo, ma la Costituzione va applicata con raziocinio, in maniera organica, armonica. Prepariamo, modifichiamo il nostro processo in modo da affrontare anche queste situazioni: con quali regole Riina interrogherà i suoi accusatori? Con quali regole lo stupratore interrogherà la vittima? Lo farà in maniera libera, perché nel nostro codice non è previsto alcunché. Quanti testimoni potranno essere chiamati a deporre Mi viene in mente che vi è un processo, in questo periodo, che riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, un processo che ha bisogno di di tempi, da bruciare, per poi mandarlo anch'esso al macero. Quindi potrà essere chiamato a testimoniare un numero illimitato di persone. Dice Mugnai, sbagliando evidentemente: ma che andate dicendo, voi dell'opposizione! Resta la norma secondo la quale il presidente del tribunale può eliminare le liste sovrabbondanti. Collega Mugnai, io non posso adesso ricordare quali sono il gioco e gli effetti del susseguirsi delle norme nel tempo. È vero che vi è questa norma del nostro codice, ma quando voi introducete una norma speciale con la quale è prevista l'obbligatorietà, a pena a pena di nullità, dell'assunzione di tutti i testimoni che vengono presentati dall'imputato quando questi testimoni sono in riferimento a prove precedentemente assunte che si vuole confutare,

avete fatto in modo di mandarne al macero centinaia di migliaia, questa volta - ancora una volta - pur di impedire che si proceda regolarmente nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri vi inventate la storia del numero dei testimoni, numero illimitato, non controllabile. è un altro aspetto, che riguarda comunque e sempre gli interessi di una persona sola. Il giudicato, le sentenze che passano in giudicato fanno stato (certo, questo fare stato, chi se ne intende lo comprende bene, ha dei limiti). Ma prevedere che tutti i testimoni che siano stati esaminati in un precedente giudizio concluso con sentenza passata in giudicato, e delle cui dichiarazioni l'estensore della sentenza abbia fatto un uso, le abbiano tenute in considerazione, possano essere ricitati e reinterrogati, come se nulla fosse accaduto, come se nessun giudizio ci fosse stato in precedenza, anche questo mi fa pensare ad un processo in corso, in cui dà fastidio che sia intervenuta una precedente sentenza di condanna.

le ragioni per cui viene introdotta questa riforma. Qual è l'esigenza che norme di questo genere vanno a soddisfare? Vorrei comprenderlo. Secondo me non c'è un'esigenza di questo tipo, a meno che, come ho detto ieri e ribadisco oggi, non partiate tutti dall'idea che la magistratura sia un'accozzaglia di matti, sia costituita in Italia da soggetti pericolosi. Allora, colleghi, abbiate il coraggio e la coerenza di adottare norme che abroghino l'attuale magistratura,

e di cui non state tenendo minimamente in considerazione il punto di vista. Si è svolto un *referendum* che ha detto con chiarezza che cosa vuole il popolo italiano: vuole che i cittadini siano uguali davanti alla legge, vuole che si proceda nei confronti di chiunque sia stato accusato o in modo che questi sia

di tipo particolare che hanno reso l'andamento dell'attività giudiziaria a dir poco difficile, una corsa ad ostacoli. Immaginate voi l'introduzione di queste norme che cosa provocherà. Non stiamo parlando di

è responsabile il comportamento del pubblico accusatore. E non c'è bisogno di fare tante riforme, né tante modifiche, perché sarà il tempo e la volontà e la capacità di giudicare di tutti a verificare se le accuse sono sistematicamente infondate, e rispondono ad una esigenza del Paese. Mi interrogo ancora una volta sulle ragioni reali per cui una maggioranza così vasta, in cui ci sono

di assumere una posizione coerente con i principi che non sono solo i nostri, ma sono i principi della nostra storia? State mortificando il processo. Perché? A cosa servono queste norme? Voglio che qualcuno di voi si alzi e spieghi la ragione per cui voi votate norme di questo tipo che sono devastanti, per il processo e per gli interessi del Paese! È cambiato il Ministro della giustizia. Io, per natura, sono ottimista. Non dovrei avere molte speranze, per una serie di valutazioni che non spiego ora

obiettivi primari, essenziali, urgenti nell'interesse dell'amministrazione della giustizia? Il Paese ne ha bisogno. C'è un'urgenza assoluta ormai, siamo ai limiti del collasso. Oppure si deve pensare che il vostro interesse è quello di paralizzare l'attività giudiziaria? Ma non posso ritenere che questo corrisponda alla verità dei fatti. Ci deve essere un meccanismo che vi blocca, che vi condiziona. Questa norma, questa legge non serve a nulla, se non a complicare ulteriormente la situazione, a rendere ancora più difficile l'attività giudiziaria e a privarci delle risposte giudiziarie delle risposte giudiziarie di cui abbiamo bisogno per sapere se una persona accusata, chiunque essa sia, è veramente responsabile o è soltanto raggiunta da un'accusa che può essere infondata. Ma saperlo in tempi rapidi è indispensabile. Saperlo dopo dieci anni vale a poco, spesso vale soltanto a inasprire ulteriormente gli animi. Quindi, su questo terreno non vedo che cosa renda impossibile un'intesa, visto che la legislatura, nonostante tutto, prosegue. Io vi chiedo di ragionare, a partire dal momento in cui andrete a decidere e a votare su questa norma, questa norma va modificata, vanno stralciate queste ipotesi assurde e dannose, che non rendono assolutamente vantaggi al Paese: potrebbero renderli ancora una volta (ma vedrete che poi, alla fine, non ci sarà questo effetto sperato) alla posizione del Presidente del Consiglio dei ministri, ma non passerà neppure questa norma, perché è visibilmente e chiaramente contraria ai principi costituzionali. Per questo, mi auguro che, almeno davanti a queste evidenti storture, a questi evidenti danni e pericoli per il Paese, possiate ragionare, e quindi interrompere questa corsa allo sfascio

soprattutto aleggia un senso di incredulità: si sta ragionando di un provvedimento di questa natura nel momento in cui il Paese è sottoposto ad una serratissima offensiva speculativa che rischia di mettere in crisi tutto il nostro assetto economico, con la forza produttiva del Paese già messa in crisi da tempo da dismissioni, dislocazioni all'estero, mancanza di lavoro per i giovani, predominio del lavoro precario e insorgenza - sono costretto a richiamare questo tema sempre più preoccupante - del lavoro gratuito, che sta diventando la categoria principale attraverso cui i giovani entrano nel mondo del lavoro. L'incredulità domina di fronte ad una atmosfera di questo tipo, che è riassunta del Presidente del Consiglio nel momento in cui finalmente sostituisce il Ministro della giustizia. Appare chiaro che il suo obiettivo principale è quello che lui dice al suo Ministro (da notare l'espressione vagamente padronale): «Tu devi fare la separazione delle carriere»; e il Ministro, obbediente, gli risponde: «Sì, sì, farò senz'altro così». Ecco, di fronte a una crisi economica di natura impressionante, la massima preoccupazione del Presidente del Consiglio è la separazione delle carriere dei magistrati. Il chiodo fisso nella sua mente è la preoccupazione per la giustizia, e la maggioranza gli appronta uno strumento che, se fossimo dentro una narrazione di tipo immaginario, risulterebbe incredibile. Un provvedimento che ha un titolo che riguarda

un accrocco ingegneristico che introduce al suo interno il necessario per rendere privo di significato il titolo e rivolgere la legge a ben altri fini. Molti colleghi esperti di materie giuridiche si sono dilungati e ci hanno spiegato il come e il il come e il quanto di tale stravolgimento; ci hanno spiegato che si può arrivare a rifare l'istruttoria in un procedimento in corso, che le liste testimoniali possono essere allungate all'infinito; ci hanno infine sintetizzato lo stato delle cose con una formula icastica: si produce il processo lunghissimo, lo si combina con la prescrizione brevissima, e si arriva ad una sorta di demolizione del processo penale. Questo tipo di direzione e questa intenzione non hanno nessuna ragione dal punto di vista del valore generale della legge: perché mai, in una situazione in cui i processi sono già troppo lenti, si dovrebbe costruire un dispositivo per allungarli ancora di più e renderli alla fine impossibili? Perché si dovrebbe impacciare ciò che è già impacciato e invischiato in lentezze e in elementi da superare? C'è veramente qualcosa di incredibile. Dentro questo tipo di volontà c'è anche la produzione di una nuova dimensione di giustizia di classe. Voglio usare questo termine proprio specificatamente nella sua accezione storica: la giustizia di classe funziona in maniera diversa per i ricchi e per i poveri, perché è facilissimo immaginare schiere di avvocati agguerritissimi, di studi molto preparati, mettersi al servizio di un cliente facoltoso, producendo liste testimoniali lunghissime puntando al rifacimento del processo tramite la revisione delle prove; però, è difficilissimo immaginare l'imputato debole e privo di mezzi economici riuscire a produrre un sia pur minimo sforzo in questa direzione. quindi, la demolizione del processo penale e la costruzione di una nuova dimensione di giustizia di classe: la giustizia per chi può e la giustizia per chi non può. Non c'è nessuna motivazione di carattere generale; ce n'é solo una di carattere molto particolare. Gli emendamenti specifici che sottopongono a questa torsione irrimediabile il provvedimento originario sono in un certo senso firmati, si capisce a cosa servono. Nel processo Mills, l'avvocato Mills è stato condannato per essere stato corrotto da Berlusconi.

Qui si vuole produrre un provvedimento che impedisca la verifica della responsabilità e del ruolo di Berlusconi nella corruzione dell'avvocato Mills.

poi la vicenda Mondadori, che più chiara di così non potrebbe essere.*.* Il Presidente del Consiglio ha sottratto la casa editrice Mondadori al legittimo proprietario, e lo ha fatto tramite un evento corruttivo, il cui responsabile è stato accertato nella persona dell'avvocato onorevole Previti, il quale è stato condannato per questo motivo. *(Commenti del senatore Divina).* Berlusconi è l'utilizzatore finale di molteplici e ripetuti episodi di corruzione in fatti giudiziari. Quello della Mondadori è anche arrivato al suo esito finale: Berlusconi ha dovuto pagare 560 milioni per risarcire l'editore originario, che era stato privato della sua casa editrice. Stiamo assistendo a qualcosa che non è più nemmeno grottesca, perché è al di là dei limiti dell'immaginazione letteraria. letteraria. Vale la pena, per salvare il Presidente del Consiglio coinvolto in numerosi fatti di natura corruttiva e in storie giudiziarie, demolire il processo penale e condannare all'inedia strutturale tutta la storia giudiziaria futura del nostro Paese? Si può pensare di bloccare i processi di centinaia di migliaia di persone soltanto per salvare

microrganismi si incistano dentro le cellule di un ospite più grande e lavorano oscuramente a sua insaputa, ne mangiano il sangue, alterano il metabolismo interno, si moltiplicano a dismisura e alla fine generano la morte dell'ospite e, morendo l'ospite, muoiono anche loro. caso abbiamo emendamenti che si annidano dentro un disegno di legge, lo modificano in senso perverso e pervertito, ne snaturano la natura e lo uccidono.

ha bocciato la legge sul legittimo impedimento in maniera tale che voi dovreste ammettere essere inequivocabile. Non volete sentire questa voce. Peggio per voi, continuate a produrre queste nefandezze, la Corte costituzionale ve le boccerà, o in ogni caso un *referendum* ve le affosserà: la vergogna sarà cancellata dalla volontà popolare.

una circostanza che ha a che fare con tutto quello che dirò nel mio intervento. Infatti, visto che con apprezzabile coerenza la prima firmataria non ha ritenuto

per evitare che la discussione si mantenga eccessivamente sul piano delle formulazioni teoriche), potremo figurare lo scenario

Immaginiamo - e non facciamo un grandissimo sforzo di fantasia - una banda di pericolosi rapinatori, magari provenienti da Paesi dell'Est,

Questa banda di pericolosi rapinatori, per una serie di ragioni inerenti alle sue scelte imprenditoriali, decide di dedicarsi alle rapine nelle ricche ville

La banda non va troppo per il sottile (entrano, spaccano tutto, stuprano, picchiano, feriscono) e diventa il terrore della provincia di Bergamo, come di qualsiasi altra provincia del Nord, del Centro o del Sud (ma non so per quale motivo mi viene da pensare che agisca nella provincia di Bergamo). Naturalmente, scatta un'emergenza di polizia, per cui la procura, la Polizia di Stato e i Carabinieri si dedicano operosamente all'attività investigativa ad assicurare alla giustizia i componenti di questa pericolosa banda di soggetti che entrano nelle case dei bergamaschi, rapinano, stuprano e qualche volta uccidono. La Polizia, effettivamente, assieme ai Carabinieri e alla procura di Bergamo svolge un buon lavoro perché riesce a ritrovare, per esempio (succede), delle videoriprese, poiché in alcune ville erano impiantati dei sistemi di registrazione a circuito chiuso, per cui alcuni rapinatori

Insomma, per farla breve, la Polizia, a seguito di richiesta della procura della Repubblica al GIP presso il tribunale di Bergamo, arresta cinque, sei, sette rapinatori, tutti quanti individuati sulla base delle videoriprese, del rilevamento delle impronte digitali o, magari, anche del DNA che hanno lasciato sulle vittime di stupro all'interno delle ville. Nell'attuale situazione, ancorché sgangherata, della nostra legislazione processuale questi signori, se fossero consigliati da un difensore munito di un minimo di competenza professionale, di fronte a un aggregato probatorio di questo tipo chiederebbero il giudizio abbreviato. Di fronte ad una situazione normativa mutata a seguito di una legge come questa, prescindendo dalle questioni sulla ammissibilità del giudizio abbreviato (immaginiamo che non abbiano commesso omicidi, ma solo rapine, violenze e stupri), loro non chiederanno mai il giudizio abbreviato. Sarebbero pazzi a farlo, e lo sarebbero perché il processo che dovesse seguire all'arresto effettuato a seguito di una brillante operazione di polizia si svolgerebbe più o meno nel modo che vado a raccontarvi. La difesa naturalmente deve fare il suo lavoro, e il suo lavoro è, nel caso specifico, quello di tutelare i clienti, ancorché pericolosissimi e in alcuni casi rivoltanti criminali, di cercare di ottenere la loro liberazione e di farli assolvere. Ottenere la liberazione non sarà difficilissimo in relazione alla scadenza dei termini di custodia, e vi spiego rapidamente perché. Come vi ho detto all'inizio, abbiamo delle videoriprese e delle impronte digitali: questo renderebbe manifestamente superflua, per esempio, l'audizione di un gran numero di testimoni dei soggetti che si trovavano nel luogo in cui le rapine erano state commesse, anche se non li hanno mai visti in faccia (del portiere dello stabile, di chi ci faceva le pulizie, delle vittime). Immaginiamo che per dieci o cinque rapine ci siano 100 testimoni potenziali, nessuno dei quali, di fronte a un quadro probatorio come quello che ho indicato (videoregistrazioni e impronte digitali), sarebbe sarebbe necessario. La loro audizione sarebbe, per lo meno in quel numero, manifestamente superflua, ma non priva di pertinenza. Secondo la legge che voi volete approvare, tutti questi testimoni, essendo pertinenti, ancorché manifestamente superflui, dovranno essere ammessi dal giudice e, se il giudice non dovesse ammetterli, produrrebbe un provvedimento nullo, il quale farebbe cadere l'intero processo. Quindi, gli avvocati di questi rapinatori dell'Est europeo, efferati stupratori, terrore della provincia di Bergamo (collegio dell'onorevole Lussana), chiederanno 100 testimoni a difesa sulle più varie circostanze, perché, come ho cercato di ricordarvi ieri, oltre alle circostanze che hanno a che fare con il fatto reato, costituiscono oggetto di prova, e quindi oggetto di questa disciplina e oggetto di un dovere di ammissione del giudice a pena di nullità, tutte queste altre belle cose: la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo e il luogo oltre ogni altra modalità dell'azione. Se avevano delle pistole o dei mitra, la difesa potrà chiederne accurate perizie, anche se la cosa non è interessante, per verificare specificamente - si tratta di cosa manifestamente superflua ma non priva di pertinenza - il loro livello di funzionalità; potrà chiedere ogni tipo di accertamento e testimonianza, per esempio, sulle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo; potrà convocare 100 testimoni per dire che a casa è un bravo ragazzo, ama i cani e tratta bene i bambini (questa è manifestamente superflua ma non è priva di pertinenza, in relazione al combinato disposto degli articoli 187 del codice di procedura penale e 133 del codice penale). Il processo, dunque, con l'ammissione di 200 testimoni comincia in tribunali in cui - mi spiace che non ci sia

Dunque il processo comincia, e sapete come? Con l'audizione dei testi dell'accusa, magari le vittime, che i soggetti che le hanno rapinate, violentate e stuprate potranno direttamente interrogare, guardando negli occhi le persone cui

cui il tribunale non avrà alcun potere di intervento o di revoca su prove manifestamente superflue, ma pertinenti in astratto e che, in quanto tali, a seguito di questa modifica di legge, dovranno comunque obbligatoriamente essere ammesse.

che scarcerare questi assassini, rapinatori o stupratori - in ogni caso pericolosissimi criminali - i quali usciranno dal carcere e faranno marameo ai cittadini, alla giustizia a alla decenza di questo Paese.

al giudice la possibilità di decidere di filtrare e quindi di ritenere quand'è il momento di chiudere la fase del processo che riguarda l'assunzione e l'ammissibilità delle prove. Devo dire che

"e manifestamente non pertinenti salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte"».

introdotti effetti che, dal nostro punto di vista, per tutte le parti del processo (non solo l'imputato, ma anche la parte offesa o eventualmente chi si è costituito parte civile),

da dove nasce questa iniziativa, da quale dibattito culturale, da quali giuristi, in quale audizione e da chi è stata sollevata questa necessità urgente di rivedere il regime dell'ammissibilità delle prove.

*(PD)*. Anche rispetto ai contributi della dottrina e della giurisprudenza, non pare di rilevare in questi ultimi tempi

remissione tacita di querela, al trattamento previdenziale dei condannati per mafia, ai pareri del Consiglio superiore della magistratura e agli interventi a tutela della magistratura, poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, all'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale. Si potrebbe continuare con la legislazione comunitaria, cioè con tutta una lunga serie di provvedimenti di provvedimenti incardinati nel lavoro della Commissione giustizia, questi sì oggetto di audizioni, di sollecitazioni e di interlocuzioni con gli operatori e con la società civile,

importanza e una loro evidente giustificazione nell'aspirazione a riforme più complessive delle giustizia, ma per quanto riguarda un'amministrazione ordinaria, che poi non è così ordinaria. Sono tutti provvedimenti che andrebbero a incidere, a cambiare

una volta annunciati in questa Aula e ad un confronto che molte volte è pacato e costruttivo nella stessa Commissione giustizia, è davvero difficile capire come si possano introdurre modifiche di questo genere calandole all'interno di un dibattito che non aveva mai avuto il sentore né dell'urgenza né dell'importanza, tanto meno della pertinenza

fattispecie e circostanze che sono stati acclarati dentro provvedimenti e sentenze passate in giudicato debbano essere

certamente equo, ma anche tempestivo rispetto all'oggetto e alle questioni sollevate. con l'ordinamento costituzionale, ma anche nel merito, per gli effetti che produce e per il contesto nel quale matura, anche ai fini di un corretto rapporto tra maggioranza e opposizione, inserire un provvedimento che non trova alcun

le quali mi hanno formulato una pressante esigenza di poter intervenire uno per Gruppo per manifestare alcune loro obiezioni e opinioni in ordine all'avvenuta apposizione della questione di fiducia su questo disegno di legge.

Signor Presidente, ci sono delle parole che non dovrebbero essere mai pronunciate e che io faccio fatica a pronunciare,

in cui si deve usare la parola «regime», quel momento è questo. Presidente, ci troviamo in una condizione drammatica dell'Italia. Questa mattina le Borse hanno aperto in una difficoltà estrema per i nostri titoli e lo *spread* è immediatamente saltato per aria, lo Stato italiano, in questi tre anni, è stato spappolato (mi riferisco sia alla struttura dello Stato centrale che alla struttura dello Stato periferico), e noi siamo in Aula per esaminare una legge - mi dirlo - schifosa, perché mette a rischio l'intero impianto del processo penale, e lo fa - sapete che è così - per difendere gli interessi processuali di una persona che sta tenendo in ostaggio l'Italia da 15 anni

e corrompendo la testa delle persone e dei cittadini. Questa maggioranza perde

Adesso su questo provvedimento il Parlamento viene mortificato, umiliato e considerato per quello che è: un Parlamento che è stato nominato con una legge che lo stesso autore ha Presidente, noi siamo diventati un ufficio di Berlusconi e, come in tutti gli uffici, il capoufficio la mattina decide quello che il suo ufficio deve fare: che cosa deve discutere, quando deve approvare, cosa può modificare, cosa deve restare; e, se ha fretta o non vuole il dibattito, o pensa che il dibattito possa in qualche modo influire e danneggiare la sua immagine o il risultato, procede con gli strumenti che riesce a costruire: una volta armonizza e, un'altra volta, mette la fiducia. Questo è il metodo. Io non uso volentieri per il mio Paese la parola «regime», signor Presidente, ma le debbo dire che in Europa e nelle che in Europa e nelle democrazie occidentali non avremo mai un regime come quelli che abbiamo conosciuto: non avremo mai le camicie nere, le corporazioni, la marcia su Roma; noi avremo quello che stiamo avendo oggi in Italia, Italia, un sistema addomesticato e piegato nel Parlamento, che è il primo luogo che va piegato, naturalmente. Questo sta succedendo

i problemi vanno evidenziati soprattutto se gli argomenti portati in discussione hanno titoli criptici, contenuti sconosciuti e hanno anche avuto un *iter* parlamentare che il Capogruppo in quel momento presente (non ero io, ma parlo per chi era presente quel giorno) non può conoscere. Non possiamo accontentarci di un titolo che viene portato e poi per una settimana continuare a ricordare che quel calendario è stato approvato all'unanimità: non è stato approvato all'unanimità, signor C'è stato un metodo subdolo con cui la questione è stata presentata, ed è per questo che è stato approvato! Lei sa benissimo che è questo il motivo per cui è stato approvato! Lei sa benissimo che se l'opposizione fosse stata cosciente di che cosa le era stato proposto non lo avrebbe mai approvato!

signor Presidente, che lei rappresenti al Governo qual è il danno alla democrazia parlamentare che viene da questi comportamenti. questi sono comportamenti del Governo dei quali, siccome sono italiano e amo molto l'Italia, mi vergogno e che mi costringono a usare una parola che non avrei voluto usare: la parola «regime».

prendo atto con rammarico della sua lagnanza in ordine all'andamento di quella Conferenza dei Capigruppo, in relazione alla quale probabilmente vi sono state delle incomprensioni o inesatte comunicazioni. Mi faccio carico

nella loro essenzialità, nel contenuto, al di là della didascalia e del titolo. Su questo, assumo pieno e formale impegno, recependo la sua lamentela. Signor Presidente, a norma di Regolamento il Governo può mettere la fiducia quando e come ritiene. Non è questa la sede per fare valutazioni di ordine procedurale e formale (lo abbiamo già fatto ieri), quindi per brevità non ripeto le persistenti violazioni del Regolamento e della Costituzione che secondo me sono state consumate con riferimento al provvedimento

la situazione di paralisi del Paese e affermano che è necessaria una nuova manovra economica, che è necessario fare sacrifici e che già noi li abbiamo chiesti e li chiediamo alla parte più debole

così come ci ha ricordato, signor Presidente, qualche minuto fa il Capo dello Stato nel suo bellissimo intervento sul tema della giustizia organizzato dal Partito Radicale, invitandoci tutti alla coesione e al confronto sul merito delle questioni, il Governo non trova di meglio da fare che mettere la fiducia su un atto - mi consenta, signor Presidente - vile dal punto di vista politico. Si ponendo infatti la fiducia su una norma proposta dal Governo che nulla ha a che vedere con il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che è parte del disegno di legge governativo sulla riforma del processo penale, su cui, in maniera proditoria, si è cercato di contingentare il dibattito, di strozzare ogni forma di discussione, di farla passare per una banalità, di ricattare politicamente la Lega prevedendo subito dopo questo

so quanto a lei stia a cuore il sistema delle garanzie parlamentari. Questa di oggi è un'offesa: è il calcio dell'asino che viene dato al Parlamento, al Paese e alle istituzioni, e credo che tutto questo non lo meriti né il Paese, né il Senato, che con grande difficoltà ha sempre tenuto un atteggiamento di grande civiltà e di grande tolleranza anche rispetto a provvedimenti assolutamente non condivisibili. Ci consenta quindi non uno sfogo, ma una protesta. Siamo ormai disarmati di fronte a questo modo irresponsabile, inconcludente,

Presidente, si dice spesso che c'è un accrescimento della distanza tra la politica, le le istituzioni e l'Italia reale. e qui raccolgo sia l'espressione del collega Zanda, sia quella del collega D'Alia - di un fine regime, eccola in quest'Aula stamattina. L'Italia si sta interrogando sui numeri reali dell'economia. Abbiamo visto cosa sta accadendo in queste ore con l'asta dei titoli di Stato che denota un grave calo di attenzione e d'interesse degli investitori sul nostro Paese, un accrescimento degli oneri che già di per sé, signor Presidente, comporta l'adozione di un'altra manovra. E il rinvio dell'asta prevista in agosto sottintende proprio questo: il desiderio, da parte dell'attuale Ministro dell'economia, di non mettere i numeri di fronte all'evidenza della realtà e aspettare settembre.

basta alle contrapposizioni in materia di giustizia, si pone la questione di fiducia sull'ennesima legge *ad personam* e sull'ennesimo stravolgimento delle procedure del processo italiano a beneficio, di nuovo, dell'idea di risolvere o allontanare una problematica giudiziaria che riguarda il Presidente del Consiglio. Ma ci rendiamo conto che tutto ciò che accade fuori di qui non ha nulla a che vedere con ciò che si pone stamattina

una serie di interventi dei rappresentanti delle opposizioni senza che si alzi una persona dai banchi della maggioranza per dire che non è d'accordo debbo dire che lo considero

perché, con ogni probabilità, troverà uno stop dal punto di vista costituzionale e giurisdizionale, senza voler chiamare in causa le alte magistrature della Repubblica, che hanno la loro perfetta autonomia. Ma di cosa stiamo parlando?

Le opposizioni hanno consentito innanzitutto di approvare in tre giorni una manovra molto impegnativa da parte del Governo, fatto e prova di responsabilità senza precedenti.

Però siamo consapevoli che quel dibattito, colleghi, è iniziato con una dichiarazione del vice ministro Castelli che aveva detto che non avrebbe votato

drammatico delle difficoltà in cui si trova il Paese: è un elemento di autenticità. Ci sono difficoltà che coinvolgono tutti, ma le opposizioni non si tirano indietro, con le loro diversità interne, di profilo politico e anche di prospettiva. Nel momento in cui c'è da votare una manovra in 72 ore, danno il loro assenso perché ciò avvenga. Rendiamoci conto di che cosa sta accadendo in questo momento nel Congresso degli Stati Uniti, dove per

di cui continuiamo a non condividere l'ispirazione, poiché insufficiente per la crescita e inadeguata nella scelta dei tagli della spesa pubblica, pur se avremmo avuto buon gioco a inchiodarvi a queste difficoltà, tuttavia non lo abbiamo fatto.

date uno schiaffo al Parlamento, impedite persino che si parli per opporsi a questo provvedimento e ci chiedete il voto di fiducia? E poi tornerete domani a chiederci responsabilità sull'economia? Responsabilità sulla politica estera? Responsabilità sulle prospettive di questo Paese?

mettiamo le priorità al giusto posto»? Le priorità sono certamente l'economia, il decreto rimpatri - se si vuole - e le altre misure all'ordine del giorno del Senato, ma non certo l'ennesima leggina che stravolge il processo penale in Italia per l'interesse di qualcuno!

Presidente, colleghi, il colore rosso di quest'Aula è visibilmente stampato sulla faccia e nelle menti dei componenti della maggioranza. *(Applausi dal È un rosso-vergogna, senatore Centaro, se un parlamentare di vaglia come lei, con una carriera...

il senatore Centaro ha avuto persino perplessità a svolgere la relazione introduttiva in quest'Aula: questo la dice lunga, rimane addirittura fuori dalla porta, per non metterci la faccia, o meglio, per non metterci la faccia in questa maniera!

La vogliamo definire banditesca? La vogliamo definire di regime? La vogliamo definire fascista? Noi stiamo usando questi aggettivi almeno da un paio d'anni, nel silenzio di tanti e tanti, in questo Paese: alla fine, però, chi la dura la vince. Non noi, perché è il Paese che ne esce sconfitto: vincono l'arroganza, la protervia, la prepotenza l'offesa agli organi democratici. Signor Presidente del Senato, pur con il riguardo che nutro nei confronti della sua persona, non posso non evidenziare le sue dichiarazioni di questa mattina: occorre rendere più spedito il processo, ha detto il Presidente del Senato qualche ora fa. Certo, renderlo spedito allungandolo fino in fondo, ma qui non siamo dei deficienti: queste cose le capiamo, e le capiscono anche gli italiani. allora, la domanda è: quali garanzie restano al Parlamento repubblicano? costretto ad approvare in tutta fretta, mentre quella poca gente che può è in vacanza, un disegno di legge del genere? Un disegno di legge emendato,

questo è il rispetto dell'Aula? Secondo lei, che a ogni piè sospinto dice di essere garante dell'Assemblea, questa è garanzia per il Parlamento? No, signor Presidente del Senato, non è assolutamente garanzia del Parlamento.

come noi, dei termini puntuali, rigorosi, precisi, perché non è più tempo di bugie, colleghi di maggioranza.

In un momento di orgoglio, fate ammenda di quella che è un'offesa per l'intero Parlamento italiano, il che significherebbe poco, visto come ci considera il Paese: ma è un'offesa all'intero Paese e all'intera Repubblica italiana! Presidente, la storia di questo provvedimento è cominciata male ed è finita peggio. Ho avvertito più volte il suo impegno a ricondurre la vicenda entro canoni di correttezza parlamentare, ma ho anche notato il suo imbarazzo, perché è vero dal punto di vista formale nulla si può contestare. Non voglio tornare indietro, ma l'antefatto è il fondamento di questa vicenda. L'approvazione di quel calendario in Conferenza dei Capigruppo, formalmente incontestabile, si inserisce in quella previsione italiana di formalismo giuridico un po' leguleio in cui la forma fa torto alla sostanza. Oggi anche il comportamento del Governo è incontestabile. Ha tutto il diritto di porre la questione di fiducia e nel momento che preferisce, ma questa scelta, all'interno di questa vicenda, segna un *vulnus* nei rapporti parlamentari tra maggioranza e opposizione e con il Governo. Credo che questo sia davvero un grande errore politico, per la condizione drammatica del Paese, che avrebbe avuto bisogno di quell'inizio di ravvedimento operoso cercato e sollecitato dal Capo dello Stato. E' imbarazzante, e in qualche modo surreale, che, mentre a pochi metri da noi il Presidente della Repubblica sollecita una visione comune del processo riformatore inserendolo nel processo avviato sulla manovra di stabilità finanziaria, il Governo e la maggioranza, con una distonia incredibile, cerchino di varare un provvedimento imbarazzante. È imbarazzante certamente per il suo contenuto gretto per la mancanza di respiro: nessuno può nascondersi dietro l'ipocrisia di un provvedimento generale e astratto, perché si tratta di un provvedimento concreto e specifico che riguarda una fattispecie specifica, personale, che modifica e distorce il sistema processuale italiano per l'ennesima volta. Ieri la collega Della Monica, in un ammirabile intervento, oltre che contestare nel merito questo provvedimento, ha ripercorso tutte le tappe, tutti gli interventi distorsivi del nostro sistema processuale per inseguire le vicende personali, e certamente politiche, del Capo del Governo. Presidente, ho un altro rammarico. Comincia male la sua avventura una persona che stimo come il nuovo Ministro della giustizia. Qualche mese fa il ministro Alfano preannunciò una grande stagione riformatrice e l'abbandono delle leggi *ad personam*. L'area politica del Terzo Polo disse che, se questo fosse stato davvero il canovaccio di quell'azione politica, ci avrebbe trovato disponibili al dialogo e al confronto, perché a tutti interessa il ruolo della giustizia. Oggi il nuovo Ministro della giustizia annuncia il medesimo percorso e il Governo fa violenza al Parlamento con la richiesta di voto di fiducia su un provvedimento *ad personam*. Credo che abbia davvero ragione il mio collega D'Alia: questo Governo deve soltanto dimettersi.

nel calendario prima della pausa estiva. Li ricordo. Abbiamo da affrontare un importante dibattito sul bilancio del Senato, nel corso del quale andremo ad operare tagli importanti ai costi della politica, quei tagli che ci chiedono giustamente i cittadini,

Dobbiamo anche affrontare, Presidente, un importante decreto sull'immigrazione. Voglio ricordare ai colleghi dell'opposizione,

non vogliamo rimanere fermi su questo provvedimento fino alla prossima settimana. Non solo, Presidente. Credo che le opposizioni possano in questi momenti dire quello che vogliono - è giusto, e comprendiamo anche le strumentalizzazioni del caso

noi stiamo semplicemente rispettando il Regolamento. Vogliamo approvare tutti i punti all'ordine del giorno e, usando il Regolamento nel rispetto delle regole, siamo convinti di poterlo fare.

ha sempre espresso le proprie posizioni e si è sempre assunto le proprie responsabilità. Lo fa anche in questa occasione. Affinché resti a verbale del Senato, voglio anch'io, come ha fatto poc'anzi il collega Bricolo, sottolineare in primo luogo gli aspetti di natura procedurale.

farà precedere le Conferenze dei Capigruppo da un'informazione formale ai Gruppi sugli argomenti in discussione. Ma tutto questo era già avvenuto nella discussione

Ho letto articoli che descrivevano questo provvedimento come in grado di ostacolare processi per mafia. Non è vero. Ci sono colleghi che l'hanno detto in questi giorni. Il relatore e il capogruppo Mugnai hanno dimostrato, richiamando articoli citati nel disegno di legge, come tutte le attività processuali che colpiscono la criminalità organizzata non ricevono alcun nocumento. Lo dico forte di una maggioranza che su questi temi del contrasto alla criminalità - dalle leggi antimafia al 41-*bis* - ha una credibilità di gran lunga superiore a quella del vostro schieramento e delle vostre icone, che hanno fatto delle

di mentire. GASPARRI *(PdL)*. Questo è ampiamente consentito dalle norme che restano in vigore dopo l'eventuale approvazione di questa legge. Certo, si affermano alcuni principi di buon diritto. Se un imputato si vede spiattellare accuse da un altro giudizio in cui non era presente, la possibilità di verificare queste accuse è un pieno diritto di qualsiasi persona in questo Paese, per accertare in maniera trasparente le verità giudiziarie *(Applausi dal Gruppo PdL)* e non subire condanne in base a giudizi

i principi dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, che sono ripresi letteralmente, e fare una legge che si ispira alla Costituzione è un atto altissimo di civiltà giuridica e legislativa, lo rivendichiamo con trasparenza.

il fatto che ieri, a fronte di un emendamento aggiuntivo del relatore che afferma principi di severità che il nostro Gruppo, il presidente Bricolo e anche molti di voi avevano evocato,

Certamente si può fare, può rientrare nella lotta politica, in un confronto aspro, ma a fronte dell'ostruzionismo c'è la possibilità, ad esempio, di contingentare la discussione, e avete ieri rifiutato anche questa possibilità. L'armonizzazione dei tempi era stata da me richiesta e accolta come ipotesi dal Presidente del Senato poi è stata annunciata e avete detto che non andava bene, è stato rivisto questo orientamento e si è continuato con una pratica ostruzionistica a fronte della quale abbiamo diritto di decidere. Ha detto ieri il senatore Zanda: vogliamo impedire l'approvazione di questa legge. Noi vogliamo consentire l'approvazione di questa legge,

cui si ispira sono giusti: li rivendichiamo e li difendiamo con convinzione.

che è un po' pretestuoso utilizzare questa circostanza per chiamare in causa il Presidente del Senato, che ritengo abbia sempre garantito il rispetto dell'Assemblea e del ruolo della maggioranza come dell'opposizione. mentre credo sia giusto e doveroso chiamare in causa la responsabilità politica del Governo e della maggioranza che lo sostiene. È un dovere un dovere politico da parte dell'opposizione, che però, quando assume alcuni toni e accenti, determina inevitabilmente la fuoriuscita dalla dialettica parlamentare e dalla contrapposizione maggioranza-opposizione

Lo voglio dire al senatore Zanda, che apprezzo e stimo: è sbagliato politicamente dire che questo è un regime e che viviamo dentro un regime. La verità è un'altra, e fatemela dire, almeno per quanto mi riguarda e ci riguarda. Guardate, quello che a volte è insopportabile - e lo dico senza ipocrisia - è la pretesa pedagogica della sinistra di interpretare il buono, il giusto e il meglio. Non è così! Non è così: stiamo dentro contraddizioni, ma non di un regime, che non c'è in questo Paese,

dell'anomalia italiana, che continua e che persiste e della quale, senza ipocrisia, dobbiamo prendere atto. L'anomalia italiana è intrisa di berlusconismo e di antiberlusconismo viscerale, e di alcuni nodi e questioni

non affrontiamo le questioni che abbiamo di fronte con onestà intellettuale e con reciproca assunzione di responsabilità. Il Parlamento

quell'anomalia che vorrei ricordare da ultimo al senatore Rutelli. Caro Rutelli, ricorda, quando stavi da un'altra parte, che hai fatto parte di Governi dove l'opposizione - maggioranza di oggi - si è assunta la responsabilità dell'interesse nazionale quando non vi era una maggioranza in grado di garantirlo. Quindi, nella memoria e nella storia di questo Paese, ci sono le responsabilità di tutti, e faremmo bene tutti ad assumerci reciprocamente le responsabilità, di ieri e di oggi, per il domani.

Colleghi, la seduta è ripresa. La Conferenza dei Capigruppo ha deliberato quanto segue: oggi, alle ore 15,30, in via del tutto eccezionale, con l'unanimità di tutti i Capigruppo, si terrà ugualmente l'informativa del ministro Matteoli;

Il Senato poi tornerà a riunirsi lunedì pomeriggio, secondo il calendario già approvato.